nella vita ho molto colpe, ma questa non ce l'ho. PRESIDENTE. Prendiamo atto della dichiarazione del presidente Andreotti.

anche momenti di dibattito intenso che mi pare non siano ben rappresentati nel processo verbale testé letto.

Il problema allora è cosa fa il Presidente del Senato in queste ore per garantire che il Senato non riceva uno schiaffo che ritengo intollerabile

perché è un dato assolutamente rilevante che - ripeto - non è soltanto politico ma entra sul piano più elevato dei rapporti tra le istituzioni. Questo è il dato che vorrei significarle e vorrei capire da lei come possiamo andare avanti nel prosieguo dei nostri lavori, soprattutto alla luce di queste considerazioni

almeno tentando di darne una interpretazione autentica. Fui io l'autore della proposta di ieri in ordine al dibattito che si chiedeva si tenesse nel pomeriggio di domani sulla vicenda Telecom, con l'invito al Presidente del Consiglio a partecipare ai lavori. Ritenevo e ritengo di essere stato chiaro: non avevamo dato il nostro assenso al calendario che prevedeva la disponibilità del Presidente del Consiglio a riferire ad uno dei due rami del Parlamento - non sapevamo quale - nella giornata del 28 giornata del 28 settembre e ci siamo riservati il nostro diritto sacrosanto, del quale si è avvalsa l'opposizione correttamente in cinque anni della precedente legislatura, di votare in Aula le nostre proposte per fare in modo che esse venissero consacrate ed inserite nel calendario dei lavori. Abbiamo esercitato un diritto, signor Presidente, che fino a prova contraria è sancito e garantito dal nostro Regolamento. Regolamento. Sono molto amareggiato - mi creda, non tanto personalmente quanto politicamente - quando ieri sera io ed altri colleghi dell'opposizione abbiamo letto le dichiarazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento e della capogruppo Anna Finocchiaro.

si è lasciato andare alle seguenti dichiarazioni. Dopo un voto sacrosanto, correttamente e regolarmente da lei gestito, risponde: a questo punto, preso atto del voto del Senato, è evidente che l'informativa del presidente del Consiglio Romano Prodi si terrà inevitabilmente presso la Camera dei deputati. Questa è la risposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento al Senato, che si era espresso in una logica diversa. Quindi, mentre qui si esercita un atto democratico, per il Ministro per i rapporti con il Parlamento la democrazia è dare uno schiaffo alla stessa democrazia! Complimenti. Mi complimento. Analoga e maggiore amarezza

chiedere l'approvazione di un calendario dei lavori - cosa che, ripeto, quando eravate all'opposizione avevate sistematicamente chiesto - è compiere un capolavoro? Piuttosto è esercitare un sacrosanto diritto che, fino a quando siamo in democrazia, va tutelato.

maggioranza ha già privato il Senato della funzione legislativa - ricorrendo sistematicamente al voto di fiducia e spogliando i singoli parlamentari della stessa maggioranza della possibilità di partecipare al processo legislativo volete anche impedirci di fare ciò, dichiarando che è far guerra esercitare il diritto sacrosanto di chiedere la modifica del calendario con un voto? Questa è la vostra visione di democrazia? guerra guerreggiata, signor Presidente. Non credo che qui si sia fatta una guerra. Abbiamo votato, abbiamo premuto un pulsante, abbiamo fatto accendere le luci, abbiamo esercitato una delle funzioni della nostra beneamata democrazia, ovvero il diritto di voto, e quando si vota c'è libertà, colleghi della maggioranza: ricordiamolo. ricordiamolo. Quindi, l'atteggiamento sarebbe stato quello della guerra guerreggiata, con il risultato - ecco lo schiaffo, signor Presidente - che «il Governo verrà a riferire al Senato, ma si radicherà la scelta del presidente Prodi di andare alla Camera».

Ieri credevo e credo di essere stato chiaro. Il Senato attende domani pomeriggio il Presidente del Consiglio: lo attende, lo ha invitato e ha esercitato una facoltà prevista dall'articolo 59 del nostro Regolamento che recita: «I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte del Senato,» - e il Presidente del Consiglio non è senatore «hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni». Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di partecipare domani pomeriggio: secondo noi e secondo il Regolamento, che ancora è vigente, fino a quando non verrà modificato a colpi di maggioranza - ma noi ci riserviamo di esercitare il nostro diritto sacrosanto di opporci Ovvero il Presidente del Consiglio, se non vuole violare ulteriormente le regole della democrazia, offendendo il Senato, e se vuole rispettare il nostro Regolamento, ha l'obbligo sacrosanto di venire domani pomeriggio in Senato e partecipare alla seduta in occasione della quale si discuterà della vicenda Telecom. Credo che con la pacatezza con cui ieri abbiamo svolto i lavori e abbiamo preso le decisioni a cui i due interventi si sono riferiti,

cercare di rendere chiara, in questo momento, la questione che si è posta: è evidente che il presidente del Consiglio Prodi non aveva intenzione di riferire nulla, né alla Camera dei deputati

Non mi meraviglio che questo possa accadere, ma è bene che il Presidente del Senato recepisca, nel voto di ieri, la richiesta dell'opposizione di contare. Il Presidente del Consiglio

può bastare un voto, ma delle questioni della vita quotidiana, sulle quali può non bastare un voto di maggioranza. Questa è la situazione che ieri è esplosa, che rimane qualunque sia la vostra decisione, e che rende evidente che in quest'Aula

forse non farebbe male a venire qui domani pomeriggio. Sarebbe molto più serio se venisse qui. La questione sarebbe conclusa, e lui non rimarrebbe per otto giorni in attesa, senza sapere cosa dire. Fateglielo capire, ammesso che vogliate aiutarlo.

ha chiesto esplicitamente la presenza del Presidente del Consiglio al Senato nel corso della discussione prevista per domani pomeriggio.

che questa Camera, il Senato della Repubblica, non può accettare il balletto delle dichiarazioni del Governo e di qualsiasi altra fonte di opinione del nostro Paese. a mio parere, può ripristinare una legalità non solo politica, ma anche istituzionale dopo questo strappo alla democrazia. Non possiamo accettare che il Presidente del Consiglio faccia decidere tra i due Presidenti

Questo è il Senato della Repubblica; è la sede del popolo sovrano! Cari colleghi, se non facciamo rispettare queste basi

è molto saltuaria, ma oggi evidentemente è chiamato a dare il suo parere ed il suo voto su un tema notevolmente rilevante come quello dell'ordinamento giudiziario) di un senatore a vita che è stato anche Presidente della Repubblica.

i nostri predecessori senatori ebbero ad introdurre nel Regolamento. Tale articolo prevede che «i membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute». Allora, senatore Ciampi, lei è stato Presidente della Repubblica, garante della Costituzione, ha garantito il rispetto della Carta costituzionale e lo ha fatto bene: tutti gliene siamo grati e tutto il Paese lo ha riconosciuto. - ripeto - da chi è stato Presidente della Repubblica. Salutiamo con piacere l'ingresso in Aula del presidente Cossiga, anch'egli ex Capo dello Stato e quindi anch'egli autorevole e prestigioso garante del rispetto della Costituzione.

che ritengo occorra evitare per rispetto dell'unità del Paese e delle regole nelle quali tutti cittadini italiani si sentono unanimemente riconosciuti e tutelati.

*(LNP)*. Signor Presidente, poco fa lei ha accennato all'eventuale difficoltà di mettersi in collegamento telefonico con il Presidente del Consiglio. Poiché mi risulta che il contratto base del Senato e del Governo sia un contratto Telecom, suggerirei Questori di acquistare una scheda telefonica, anche una tessera a scalare, di un'altra compagnia, per aumentare la possibilità di riuscire a parlare in diretta con il Presidente del Consiglio, che evidentemente si trova su un'altra galassia e con il quale credo sia doveroso che il Presidente del Senato riesca a parlare per sapere se verrà giovedì pomeriggio, cioè domani, a riferire su una questione tanto importante come il caso Telecom. Non vorrei che la Telecom, essendo coinvolta, abbia tagliato i fili dei collegamenti con il Presidente del Consiglio.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 635.

per l'inversione dell'ordine del giorno o per l'inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno sono diverse e che sono anche richieste maggioranze diverse. Il motivo è che quando all'ordine del giorno non figura un argomento è più che giusto e fondato che sia il Senato a deliberare con maggioranze altissime nel momento in cui il Presidente lo riterrà opportuno. Al contrario, nel caso in cui l'argomento sia già

tenute separate proprio in considerazione di ciò. La situazione che oggi abbiamo di fronte è nuova, ma secondo me va risolta nel senso prospettato dai colleghi che hanno chiesto l'inversione dell'ordine del giorno.

si fa riferimento a due sedute, la n. 34 e la n. 35. Vorrei che lei chiarisse, al fine di una corretta valutazione della richiesta di inversione dell'ordine del giorno,

di ventiquattr'ore, con scansioni mattutine e pomeridiane. La scansione dell'ordine del giorno di oggi indica due temi, due temi, entrambi all'ordine del giorno dell'intera giornata e che possono essere fungibilmente sostituiti l'uno dall'altro. L'ordine del giorno è unico, la giornata è unica. è unica. I tempi sono diversi, ma viene inserita in questa fase una valutazione che spetta all'Assemblea decidere in quale ordine vada affrontata. Ho detto questo e ho salvato l'anima mia.

necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti...»: addirittura, la maggioranza, se non vuole far passare questa proposta, è tranquillissima da questo punto di vista, anche se non ne capisco la convenienza. proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o da otto Senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno.ۛ» Dunque, il Regolamento non dice che è il Presidente a decidere il quando. Aggiunge che: «Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la Commissione può riferire oralmente». Presidente, lei ha l'obbligo di mettere in discussione e in votazione la proposta di

poiché stiamo discutendo un problema di opportunità e di approfondimento della questione, dinanzi alla richiesta formale che è stata presentata

Questa è la richiesta e la metterò ai voti, in base all'articolo 56 del Regolamento, richiamato esplicitamente dal senatore

è questione assolutamente rilevante e importante per la finanza del Paese e per la correttezza istituzionale del comportamento del fisco italiano nei confronti dei contribuenti. Come già è stato argomentato anche poco fa, nell'acceso dibattito relativo al necessario, opportuno e prossimo intervento del Presidente del Consiglio sulla vicenda Telecom, vicenda Telecom, devo constatare che la sospensiva dei decreti legislativi in materia di ordine giudiziario non possa essere considerata così urgente come invece lo è la discussione dei due argomenti Telecom e IVA,

L'importanza sta nella consistenza finanziaria che consegue la deliberazione della Corte dell'Unione Europea.

questa disavventura - chiamiamola così - causa dell'inazione del precedente Governo (ma ne discuteremo quando entreremo nel merito della discussione generale del provvedimento). Mi sembra, invece, di dover constatare, come tutti sappiamo, che anni di una normativa oggi definita illegittima, dall'Unione Europea, definita a suo tempo provvisoria (ma come sappiamo nel nostro Paese spesso ciò che è provvisorio è molto più definitivo del definitivo), sia necessario

diritti e possa tornare in possesso dei denari che la fiscalità del Paese gli ha indebitamente sottratto per tanti anni.

necessità di predisporre una legge finanziaria volta tanto alla crescita e allo sviluppo, quanto al controllo e al rientro del debito pubblico e della spesa pubblica,

di un'ulteriore riduzione di tali cifre, a fronte anche di una nuova entrata fiscale nei primi mesi dell'anno che ha mostrato incrementi indubbiamente consistenti. Tali incrementi, a mio avviso, sono dovuti all'azione - al contrario di quanto invece sosteneva il vice ministro Visco - molto puntuale di riduzione del carico fiscale, effettuata durante la scorsa legislatura. Parlare quindi, in questo contesto, di un decreto-legge che mette in chiaro le condizioni di attuazione della delibera della Corte di giustizia delle Comunità europee

entro fine mese, presentare il disegno di legge finanziaria con le modifiche alla legge del bilancio dello Stato per l'anno prossimo, quindi per il 2007, tenendo conto delle soluzioni, anche in

tornare in auge cifre sul cuneo fiscale, sulla distribuzione all'interno delle categorie impresa e lavoratori interessati di percentuali diverse di assegnazione di benefìci. Parliamo di un cuneo fiscale che può valere 10, 11 o 12 miliardi di euro; parliamo di una riduzione, di un rimborso di importi IVA indebitamente percepiti negli ultimi tre anni di 10 miliardi di euro. Signori, penso che davvero, avvicinandosi a passi lesti il periodo della sessione di bilancio, sia assolutamente necessario

che ha leso i loro diritti sostanziali, i loro bilanci, la redditività delle loro aziende, imponendo misure diverse a seconda dei tempi. Ricordavo

all'applicazione di una sentenza europea che ristabilisce finalmente - purtroppo non riusciamo a farlo in questo Paese e dobbiamo essere costretti dall'Unione Europea - diritti

La Costituzione stessa prevede che entro cinque giorni il decreto-legge sia presentato alle Camere. La 1a Commissione nella seduta di ieri ha tempestivamente esaminato i presupposti costituzionali e,

era estremamente importante ed è stato riconosciuto fondato anche dal relatore che, come di norma, appartiene alla maggioranza. Il rilievo consisteva nel fatto che esiste una sentenza della una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che ha ritenuto illegittimo e non conforme alle norme europee il regime di non detraibilità a cui sono sottoposte certe spese nella nostra legislazione. Questo decreto-legge non interverrebbe sulle norme che la Corte ha ritenuto non conformi al diritto europeo, limitandosi ad un intervento riguardante la possibilità di chiedere il rimborso. troviamo, pertanto, in una situazione in cui si può chiedere il rimborso per una detrazione di cui non si è potuto fruire perché le norme italiane ne impedivano la fruizione, ma si continua a ritenere non detraibile quella spesa per la quale pure si può chiedere il rimborso.

legislatura abbiamo approvato all'ordinamento giudiziario italiano. Anche su questo ci sarebbe parecchio da dire e sicuramente lo si se vi è una cosa su cui tutti concordano è che l'ordinamento giudiziario attuale abbia degli enormi problemi, uno dei quali - torniamo ai problemi delle imprese - è che nel nostro Paese per ottenere giustizia

che cerca di reintrodurre la certezza e la velocizzazione del diritto? Avere ragione in una causa civile - figuriamoci penale - dopo un tempo irragionevole è come non avere ragione del tutto.

in una incertezza che impedisce investimenti e l'avvio di attività. Allo stesso modo il non sapere come funziona la detraibilità dell'IVA

presentato dal Governo quando il calendario è già stato approvato. Ove questo non accadesse, dovrebbe essere il Governo stesso a chiedere che il provvedimento, che ha ritenuto di prendere per un caso di straordinaria necessità ed urgenza, venga con altrettanta urgenza esaminato dal Parlamento. A questo - ricordo appunto - si aggiunge quanto ha

mossi. Se però tutti questi ragionamenti che mi paiono di buonsenso, di rispetto per la certezza del diritto, di attenzione per i problemi di coloro che in questo Paese alla fine garantiscono fine garantiscono la produzione della ricchezza, il sostentamento delle istituzioni, siano esse del Parlamento o dell'ordinamento giudiziario; se tutto questo passa in secondo piano rispetto a considerazioni di carattere meramente di parte per cui per questioni che non hanno nulla a che fare con l'interesse dei cittadini si vuole a tutti i costi bloccare questo ordinamento giudiziario

del decreto-legge rispetto a questa controriforma, questa volta in senso veramente letterale dell'ordinamento giudiziario. Se poi la maggioranza la maggioranza e il Governo ritengono di fermare questa riforma, perché hanno ricevuto pressioni da parte di alcune componenti dell'ordine giudiziario, la questione è ancora più importante. Ovvero si tratta di sapere se le leggi debbano essere fatte - come prevede la Costituzione - dal Parlamento e all'ordinamento giudiziario spetti di applicarle fedelmente, oppure se certe

credo sia assolutamente indispensabile ricordare ai colleghi tutta la normativa che ci interessa e i motivi che sostengono la richiesta di questa urgenza, non solo nell' interesse politico delle parti che la presentano, ma soprattutto nell'interesse economico di centinaia di migliaia di imprese che aspettano questo rimborso.

in materia di «Armonizzazione della legislazione degli Stati membri relativa alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme», impone che gli Stati membri, per rispettare l'obbligo procedurale di consultazione - di cui all'articolo 29 della medesima direttiva informino il Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, istituito da tale articolo, del fatto che essi intendono adottare una misura nazionale che deroga al regime generale delle detrazioni delle imposte.

dal regime delle detrazioni di tale imposta». Ancora, al terzo comma della sentenza - naturalmente ometto le altre parti del dispositivo per ragioni di brevità qualora un'esclusione del regime delle detrazioni non sia stata stabilita conformemente all'articolo 17 numero 7 della stessa direttiva n. 77/388, le autorità tributarie nazionali non possono opporre ad un soggetto passivo una disposizione che deroga al principio del diritto delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto, enunciato appunto dall'articolo 17 numero 1 di tale direttiva. Il soggetto passivo - ripeto che si tratta di centinaia di migliaia di imprese - cui sia stata applicata tale misura derogatoria, deve poter ricalcolare il suo debito d'imposta sul valore aggiunto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, comma 2, della Sesta Direttiva 77/388, nella misura in cui i beni ed i servizi siano stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.

restituire (giustamente, in base a tale sentenza) a tutte le imprese che l'abbiano già versata dal 2000, e trovandosi quindi nell'impossibilità

abbiamo due diverse posizioni: quella del Governo, che non sa come reperire i fondi, e quella delle imprese, che invece devono prepararsi a ricevere i fondi che, indebitamente, in base alla direttiva che il Governo ha sottaciuto, hanno dovuto pagare

del rimborso dell'IRAP che adesso il Governo dovrà preoccuparsi di dare in adempimento di una sentenza di condanna, che tra qualche giorno sarà emessa nei confronti del Governo italiano, per quanto riguarda la stessa restituzione dell'IRAP, di cui abbiamo già parlato in sede di approvazione della legge

perché questa enorme massa di denaro che le imprese hanno dovuto pagare, soprattutto, rispetto all'anticipo della tassa dell'IRPEG

A differenza della Camera dei deputati, infatti, facciamo parte di un'Assemblea legislativa nella quale, seduta per seduta, mezza giornata per mezza giornata, si stabilisce il calendario

si vuole evitare che potenziali tattiche ostruzionistiche o improvvisazioni di questa o quella parte politica possano indurre disordini nello svolgimento di tali lavori. Quindi, quando si chiede di inserire all'ordine del giorno un nuovo argomento si ritiene

non ha mostrato immediatamente intelligenza politica, facendo capire che la regola dei due terzi sta proprio a dimostrare l'eccezionalità del ricorso a questa ipotesi. In questo caso la vicenda poteva essere vissuta come strumentalizzazione ostruzionistica dell'opposizione o come un'opportunità per lo svolgimento dei nostri lavori. Il motivo per il quale questa seconda considerazione avrebbe dovuto indurre

è che la razionalità dello svolgimento dei nostri lavori richiede che si voti prima sul presupposto di costituzionalità, alla luce sia della materia oggetto specifico della nostra deliberazione sia di quanto è accaduto in Commissione affari costituzionali. Se si fosse considerato questo aspetto, si sarebbe tenuto presente che in Commissione affari costituzionali l'opposizione non ha fatto tattica ostruzionistica votando contro un decreto per voler portare in Aula la questione dei cinque giorni.

È il Regolamento del Senato che considera le astensioni voti contrari. Tutto faceva presupporre che in Aula l'opposizione, se pure avesse continuato a votare astenendosi, non si sarebbe messa contro il provvedimento in maniera forte e la maggioranza - come immagino, data la presenza massiccia - sarebbe stata in grado di accettare i presupposti di costituzionalità, così come è in grado di respingere le pregiudiziali sull'ordinamento giudiziario. Intendo dire

potrebbe non esserci, quanto per l'insufficiente intelligenza politica della maggioranza. Lo dico perché si possano valutare fino in fondo casi analoghi che potrebbero capitare in futuro.

Cerchiamo di far capire ora che quella stagione si è conclusa. Non si può procedere - anche per come lei ha ripetutamente affermato nel corso delle ultime settimane - con voti di fiducia su tutti i provvedimenti. È stato possibile farlo sui decreti-legge

Ciò ha fatto sì che il partito di maggioranza relativa, il partito democristiano al Senato, avesse ripetutamente utilizzato il Regolamento parlamentare proprio per consentire la governabilità dell'Assemblea, senza irrigidirsi sul rispetto delle norme purché sia, perché questo fatto avrebbe comportato l'impossibilità di governo. Poiché i Governi della cosiddetta Prima Repubblica erano normalmente di breve durata, era essenziale che nella breve durata le Camere funzionassero. Per tali ragioni, c'è stata una battaglia durissima contro il voto segreto, vinta dopo molti anni, e c'è stata una battaglia molto seria di intelligenza politica sull'uso del Regolamento del Senato. Occorre, quindi, che la maggioranza capisca politicamente che dal 19 settembre in poi, cioè da ieri, non potrà più utilizzare le sedute antimeridiane e pomeridiane per portare avanti i suoi provvedimenti. Pensiamo a quello che succederà al provvedimento del Governo sull'ordinamento giudiziario:

noi saremo indotti a fare uso del Regolamento in modo tale da essere portati a non far funzionare il Senato. Allora, se c'è questa intelligenza, a partire dal provvedimento sull'ordinamento giudiziario o dalla questione dell'inserimento all'ordine del giorno di un punto che non era previsto per la seduta di questa mattina, se si fa capire che c'è un'urgenza condivisa su un provvedimento, non c'è ragione di utilizzare due o tre ore di discussione generale. Lo stiamo facendo e lo faremo soltanto perché la maggioranza continua nella sua ottusità

Poiché siamo ancora al 20 settembre, ho il terrore di cosa succederà da qui al mese di dicembre. Ho il terrore, con il senso di cultura del governo che mi che mi caratterizza sia per la provenienza dal partito democristiano sia per aver svolto la funzione di Capogruppo durante gli anni del Governo di centro-destra, dell'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea. Inoltre, ho il timore che si esponga il Presidente del Senato ad un'azione impropria,

parli con molta attenzione con i colleghi Capigruppo della maggioranza, cerchi di capire fino in fondo se c'è la disponibilità almeno all'intesa istituzionale, che non è l'inciucio,

Presidente, mi consentirà di rivolgermi a lei per l'attenzione che, con grande garbo, riserva sempre agli interventi in

se chiamassimo i carabinieri. Il problema di fondo qual è e perché si arriva a discutere di questo tema? Il tema che era all'ordine del giorno della seduta pomeridiana non viene posto all'attenzione dell'Assemblea da una richiesta dell'opposizione sconfitta in Commissione affari costituzionali. Faccio riferimento al Regolamento, cioè all'articolo 78, commi 3e 4:

questo caso siete obbligati ad inserire all'ordine del giorno quella deliberazione non perché l'opposizione lo abbia chiesto, ma perché la maggioranza non era in Commissione. Ha ragione il presidente D'Onofrio quando dice che la seduta della Commissione di ieri si è svolta in un clima di assoluta pacatezza. Le voglio dire, Presidente,

Governo. Prudenza vuole allora che si affronti un argomento, tutto sommato pacifico, su cui non c'è un'opposizione ostruzionistica. Ribadisco, siamo in Aula

con interventi fiume dei relatori e dei rappresentanti del Governo, perché se si azzardano a rispettare le regole vanno sempre sotto. Questo diventa allora un problema politico, signor Presidente.

o, se l'Aula deciderà di respingere imprudentemente la nostra richiesta di inserimento, poi anche sul decreto, perché, Presidente, avremo modo di discuterne.

se la maggioranza imprudentemente ha ritenuto che esistessero i requisiti di necessità e urgenza per correggere un decreto legislativo, non per correggere una norma approvata con un decreto - legge

che riguarda proprio il tema politico che ho posto, vale a dire la necessità della maggioranza di convincersi che la situazione è sempre più a rischio in quest'Aula, oltre che, come abbiamo visto, nelle Commissioni.

l'ipotesi di una discussione delle vecchie dimissioni dei senatori membri del Governo: devo dedurne che non sono state presentate. di un altro problema politico posto dal Presidente del Consiglio per far sì che l'attuale maggioranza non ballasse più. Se nemmeno quello c'è più, come fate ad andare avanti con tanta sicurezza sull'ordinamento giudiziario, sul decreto sull'IVA e su chissà quale altra diavoleria inventerete? Ecco perché le suggerisco un'iniziativa, mi scusi se mi permetto e faccio riferimento all'autorevolezza della sua carica: è il momento di far capire ai Capigruppo dell'Unione

dei presupposti di necessità e urgenza, che siamo costretti a votare perché la maggioranza è stata battuta nella Commissione competente e non per colpa dell'opposizione. sarebbe opera di saggezza da parte sua rivolgere un appello all'Unione affinché queste parole non cadano nel vuoto. Altrimenti, ognuno è causa del proprio male.

Presidente, intervengo perché rimanga agli atti il mio dissenso circa l'interpretazione del Regolamento da lei

Essi hanno sottoposto alla nostra attenzione il fatto che, quando si parla di ordine del giorno, si deve fare riferimento all'ordine del giorno di tutta tutta la giornata: non della seduta in specifico ma delle sedute previste nella giornata. Ripeto che se questa è l'interpretazione, noi avremmo dovuto applicare il comma 3 dell'articolo 56.

quando si sarebbe passati ad altro punto all' ordine del giorno e non interrompendo la discussione circa l'ordine del giorno che eravamo chiamati ad affrontare.

Senatore Ripamonti, sulla sua seconda osservazione debbo dire che noi non avevamo ripreso i lavori secondo l'ordine del giorno come non li abbiamo ripresi. Eravamo in discussione sui richiami al Regolamento quindi è stato giusto quanto fatto. Per quanto riguarda le mie osservazioni, la seduta è quella di questa mattina. Il comma quattro è estremamente preciso su questo. Lei ha la sua opinione ma io debbo ribadire la mia certezza di aver seguito il Regolamento.

una situazione a mio avviso contraddetta da una serie di elementi oggettivi. Sostanzialmente, si sostiene che dinanzi a noi è squadernato un problema politico consistente nell'impossibilità per la maggioranza di assistere il lavoro del Governo e di registrare continuamente nelle votazioni di Commissione e di Aula, appunto, la maggioranza. Vorrei fare una prima osservazione al senatore Storace, cioè che l'atteggiamento di stamattina e di ieri pomeriggio dell'opposizione sono strettamente orientati a non farci votare. Mi pare che serpeggi, anche tra le file dell'opposizione, la difficoltà e la preoccupazione per il fatto che, su voti importanti come quelli che riguardano

politica che voglio affrontare. L'assunto è che questa maggioranza non sia in grado di fare il proprio mestiere e che troppe sono le difficoltà perché questo avvenga.

ma credo che rappresenti, più complessivamente, un problema per il Senato. Nelle prime volenterose discussioni che hanno segnato l'avvio di legislatura, dal presidente Schifani e non solo sono venute, più e più volte, osservazioni che io ho totalmente condiviso e che non a caso ho ripreso nei primi interventi in Aula - che mi pare abbiano incrociato anche osservazioni fatte dal presidente D'Onofrio

Vedete, alla Camera, dove siedono *leader* politici del calibro del presidente Berlusconi, del presidente Fini e del presidente Casini, la decisione del presidente Prodi, la disponibilità mostrata nei confronti dell'invito rivoltogli dalle Camere,

diversa alla Camera, dove la maggioranza ha numeri più rilevanti ma dove siedono anche rappresentanti assai autorevoli dell'opposizione. è una cifra, nella relazione tra maggioranza e opposizione, che è centrata sul rispetto istituzionale e sulla collaborazione, ovviamente nella diversità e nel conflitto, rispetto al funzionamento delle istituzioni e alla qualità della relazione tra Parlamento e Governo. La conduzione ieri della Conferenza dei Capigruppo da parte dei colleghi dell'opposizione e poi anche gli interventi in Aula ieri e oggi, mi danno quasi l'impressione, invece, che, non nella debolezza della maggioranza,

perché riteniamo che questa Camera abbia un valore ed una importanza, nel quadro istituzionale, straordinaria e certamente non può ordinarsi gerarchicamente in nessun modo l'importanza della Camera e del Senato. STORACE *(AN)*. Dillo

perché francamente possiamo pronunciare qualunque discorso, ma che da ieri pomeriggio, in quest'Aula, l'opposizione stia lavorando costantemente perché il Senato non voti e non voti su questioni importanti come ordinamento giudiziario e decreto IVA è una costante! LNP. Richiami del Presidente)*. Noi, per quanto ci riguarda, continueremo a tentare di fare il nostro con la maggiore dignità possibile, per la maggioranza e per il Senato.

modifica delle leggi approvate sull'ordinamento giudiziario tendono proprio a ristabilire l'ordine costituzionale...

con dovizia di particolari le ragioni che rendono assolutamente singolare il disegno di legge che ci apprestiamo a discutere,

Questa è la sintesi alla quale fatalmente si è giunti. Devo dire che, contraddicendo lo spirito del disegno di legge, il Ministro della giustizia ha rappresentato quali potrebbero essere le ipotesi di lavoro che a suo avviso potrebbero migliorare il testo, legge dello Stato, che licenziammo nella scorsa legislatura. Lo strumento però adottato

un disegno di legge che chiede di sospendere ogni tipo di normativa che regolamenti l'attività, il ruolo, la funzione della magistratura italiana, perché fatalmente questo sarebbe il risultato. La legge Castelli (la chiamo così in omaggio al Ministro che ne fu promotore e che con grande determinazione si batté perché quel provvedimento giungesse a conclusione) ha abrogato una serie di norme relative all'ordinamento giudiziario. Nel momento in cui, signori dell'opposizione, si dovesse sospendere l'effetto dei decreti delegati, che sono già in corso di attuazione, non avremmo regole. Allora, appare veramente singolare, senatore Casson, che lei faccia riferimento all'articolo 97 della Costituzione invocando le massime attenzioni per la buona amministrazione, sottolineando che la Costituzione questo prevede con con l'autorevolezza che il documento comporta intrinsecamente, quando poi si sollecita una soluzione che renderebbe priva di regole, perlomeno fino al luglio 2007, al luglio 2007, la struttura di garanzia dello Stato, la magistratura. Che cosa accadrà della disciplina? Non può essere applicata la vecchia legge, signor Presidente; non può rivivere autonomamente il vecchio ordinamento giudiziario. Quali saranno le regole in forza delle quali avremo una disciplina regolamentata? Gli uffici di procura saranno affidati a chi? Alla gestione assolutamente autonoma di ogni sostituto procuratore? Quali saranno gli agganci normativi ai quali la magistratura si dovrà rivolgere per poter governare nel rispetto della legge la propria attività? Ecco il paradosso che si viene a realizzare: un vuoto normativo

non è avvenuto in maniera peregrina e che molto si può salvare. Allora, non sarebbe stato meglio, signori senatori, se ci fosse stato un testo sul quale confrontarsi? Che significato ha questa*vacatio*, questa mancanza di regole con la quale dovremo confrontarci per almeno un anno? Cosa accadrà in questo anno? E se per avventura - lo auguro, è un mio auspicio naturalmente, ma la maggioranza ha opinioni diverse - cadesse il Governo? E se si dovesse andare a nuove elezioni? E se le vicende della politica non consentissero di immaginare soluzioni alternative? Resteremmo in questo stato di limbo normativo ancora per quanto?

Ognuno di noi è qui senza vincolo di mandato e risponde alla propria coscienza e credo che la coscienza di tutti noi ci imponga di stabilire che la magistratura italiana non può andare avanti carente di regole. Per questa ragione confido che la pregiudiziale di incostituzionalità possa essere approvata dall'Assemblea. In conclusione, signor Presidente,

Ricordiamo sempre che la magistratura è una grande struttura di garanzia; una garanzia per tutti. Ed una garanzia priva di regole che cos'è?

Signor Presidente, colleghi senatori, la Lega Nord ha presentato una questione sospensiva, oltre ad una questione pregiudiziale di costituzionalità,

un vuoto legislativo nell'applicazione dei decreti legislativi a seguito della riforma dell'ordinamento giudiziario e non si intervenga invece, se lo si ritiene necessario, attraverso una modifica della legge a suo tempo approvata.

«(...) prima di approvare il provvedimento in esame, al fine di poter riscontrare la reale necessità di sospendere l'efficacia dei suddetti decreti, per un notevole lasso di tempo»; in sostanza, si ritiene il tipo di incidenza che i decreti legislativi hanno avuto nel nostro sistema giudiziario, le problematiche sollevate e i risultati raggiunti, positivi o negativi, dopo di chè si può intervenire, non tanto con una sospensione

perché tutte le funzioni costituzionalmente previste nel mondo della magistratura sono compiute;

Intervenire in questo modo è causa invece della peggiore condizione possibile per il regolare svolgimento e la chiarezza del diritto nel nostro sistema giudiziario. In discussione generale verranno indubbiamente illustrate le motivazioni tecniche e la validità delle scelte politiche per cui è stata approntata e approvata nella scorsa legislatura la riforma dell'ordinamento giudiziario. Non voglio pertanto commentare adesso le parti, i decreti legislativi e le motivazioni specifiche per cui alcuni hanno visto sospesa nella proposta del Governo la loro efficacia. Però è inutile nascondere che dietro a questo repentino, rapido desiderio di sospendere l'efficacia dei decreti applicativi più importanti è l'avversione ad una riforma del sistema giudiziario che, bene o male, discussa ma voluta comunque dalle Camere, è stato un tentativo molto profondo credo - se fosse consentito al tempo di dare le risposte opportune - anche proficuo affinché il grave limite, quello che il ministro della giustizia nella scorsa legislatura, Castelli, chiamava il debito pubblico giudiziario italiano potesse essere intaccato. In questo caso, invece, ci troviamo di fronte ad una sospensione degli effetti del lavoro svolto, a una incapacità di provvedere con proposte alternative, discutibili, sulle quali innestare un dibattito, come è stato fatto profondamente nella scorsa legislatura, con proposte alternative, che evidentemente non ci sono. Ho la netta impressione, in poche parole, che

dice che vuole tentare concretamente di dare una risposta moderna, innovatrice, riformatrice della realtà giudiziaria italiana, non lo fa certamente rinviando delle scelte operate e discusse. inutile ricordare che vi sono state varie parti in gioco, alcune delle quali ritenevano che queste scelte fossero eccessivamente profonde nella loro trasformazione, altre le ritenevano insufficienti. Dopo questa lunga discussione ci si troverà a non avere nessuna risposta concreta. Vediamo qual è la situazione nel mondo giudiziario: ebbene, non vedo oggi, anche alla lettura del programma elettorale dell'Unione, dell'Unione, soluzioni concrete, proposte che possano andare non tanto contro una riforma approvata nella scorsa legislatura, che invece è quello che si fa, ma a favore di una proposta alternativa, concreta che abbia come obiettivo il raggiungimento di una qualità della giustizia italiana che sia pari ai livelli di altri Paesi occidentali che, sotto questo profilo, non possono che definirsi più evoluti. I tempi dei processi, la situazione all'interno della magistratura, ma di tutto il mondo legato alla giustizia italiana, anche ovviamente quello degli avvocati, è gravemente in difficoltà. Si tratta di una difficoltà dovuta a un sistema giudiziario vecchio, obsoleto, che non è in grado di dare risposte. Cosa facciamo? Cosa propone invece il Governo? Propone di sospendere le riforme approvate nella scorsa legislatura,

riforme - o delle controriforme - che avranno come primo soggetto beneficiario degli interventi legislativi il cittadino e l'impresa, che oggi sono ancora e lo saranno purtroppo per lungo tempo - non dei fruitori di un servizio positivo, dinamico e rapido

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo 101 della Costituzione, che apre il titolo IV sulla magistratura, è chiaro. «La giustizia è amministrata in nome del popolo» e aggiunge: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». I due postulati sono le regole di giustizia sono scritte dal popolo attraverso i suoi rappresentanti in Parlamento e i giudici sono soggetti a queste regole. Essi sono indipendenti da ogni altro potere, ma dipendono dalla legge e dalla volontà popolare. Il giorno in cui si dovesse accettare l'idea o si avesse solo il sospetto che le leggi, ossia le regole, vengono scritte dai giudici attraverso pressioni e condizionamenti sulle forze politiche e sulle maggioranze parlamentari, si violerebbe la Costituzione formalmente e sostanzialmente. Siamo stati sempre dell'idea che non ci debbano essere invasioni di campo: liberi i giudici da condizionamenti esterni, ma liberi anche i parlamentari da condizionamenti anche da parte dell'Associazione nazionale dei magistrati. Abbiamo la sensazione che la sospensione della riforma dell'ordinamento giudiziario sia una scelta del Governo e della sua maggioranza, dettata dal sindacato delle toghe: l'opposizione forte e decisa è venuta da loro, prima che dal centro-sinistra. Questa subalternità del potere politico, le cui ragioni lascio all'immaginazione politica, ci preoccupa e ci stimola a reagire. L'UDC ha votato a favore della riforma dell'ordinamento giudiziario con senso critico e qualche perplessità, nella XIV legislatura. Il presidente Casini ha connotato tutta la sua esperienza di Presidente della Camera dei deputati all'insegna della centralità e della neutralità politica ed ha anche connotato l'immagine e l'azione dell'UDC come partito delle istituzioni, nel senso che le istituzioni democratiche devono venire prima degli interessi di potere dei partiti e delle coalizioni. Questa consapevolezza ci ha reso critici verso chiusure preconcette ed aperti ad un sano dialogo con il centro‑sinistra sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Abbiamo aperto occhi ed orecchi quando abbiamo avvertito atteggiamenti costruttivi, ma non abbiamo potuto cedere a logiche ostruzionistiche e di parte del centro-sinistra, rispetto ad una riforma che si aspettava dal 1948, ossia dall'approvazione della VII disposizione transitoria della Costituzione. La relazione del ministro Mastella, che abbiamo apprezzato per l'onestà politica con cui ha denunciato i limiti di volontà distruttive del lavoro legislativo della XIV legislatura, è un riconoscimento positivo dei fondamentali della riforma dell'ordinamento giudiziario. Il ministro Mastella ha riconosciuto infatti che la riforma è da confermare nei suoi caratteri essenziali.

Lei, ministro Mastella, ha sostenuto di volere «ricalibrare alcuni dei meccanismi posti dai decreti legislativi» realizzare questi interventi minori, chiede di sospendere l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 106, 109 e 160 del 2006, fino alla data del primo marzo del 2007. Con l'emendamento 4.0.600 del Governo, la sospensione è protratta al 31 luglio del 2007 sicché, salvaguardati gli effetti prodotti dalla riforma Castelli, dal 1° agosto del 2007 dovrebbero rivivere le disposizioni della stessa riforma.

L'unico ragionamento oggettivo, e forse convincente, è stato quello mutuato dalle considerazioni del vice presidente del Consiglio sull'ingorgo dell'attività dello stesso CSM, per l'avvio del nuovo rito sull'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Se questo è il solo problema, possiamo Se tutti gli altri istituti riguardanti l'accesso, la scuola superiore della magistratura, la separazione delle funzioni, la progressione di carriera, i concorsi, l'ufficio del procuratore e la tipizzazione degli illeciti disciplinari sono stati riconosciuti nelle valutazioni di merito da parte dello stesso Ministro come istituti da salvaguardare, salvo alcuni meccanismi di ricalibratura,

intellettuale e politica del Ministro e non intendiamo il suo discorso come un mero equilibrismo politico, bensì come un equilibrio di posizioni da raggiungere per una riscrittura di regole condivise, riteniamo che questa volontà vada colta, ma meglio esplicitata, soprattutto nel percorso legislativo di riscrittura da svolgere prima della scadenza dei termini del 29 settembre. Dobbiamo pretendere dal Ministro maggiore chiarezza ed una possibilità di percorso da poter verificare prima ancora

favorire un confronto positivo verso il quale siamo ben disposti a ragionare, come lo eravamo già nella XIV legislatura,

non si può venir meno perché è sotto gli occhi di tutti. Ebbene, questa difficoltà non può essere superata

se per la collega Finocchiaro esercitare i diritti regolamentari e il sacrosanto diritto di voto d'Aula su tutte le dinamiche parlamentari significa trasformare il Senato in un pantano, temo che la visione della democrazia della collega Finocchiaro sia estremamente preoccupante. *(Applausi Signor Presidente, ieri abbiamo votato, lei è stato il garante di quel voto e deve darci atto, come lo diamo a lei, della correttezza del reciproco comportamento. Ciascuno ha svolto la propria parte, la propria funzione,

noi non abbiamo paura del voto, signor Presidente, colleghi della maggioranza, non lo temiamo. Siete stati voi, ieri, dopo essere andati in minoranza sul calendario a fuggire dal voto sulle pregiudiziali. Presidente, ci troviamo a discutere una pregiudiziale di costituzionalità su un disegno di legge estremamente imbarazzante imbarazzante e non soltanto per il significato politico. Si tratta infatti di sospendere l'efficacia di norme prevalentemente già entrate in vigore, senza arrecare alcunché di catastrofico all'interno del sistema giudiziario. Due decreti su tre sono entrati in vigore e non si paventa alcun trauma o sconquassamento all'interno del mondo della giustizia. Ciò che imbarazza, colleghi, è leggere le motivazioni del disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia - sono atti parlamentari - allorquando si sostiene che sostanzialmente l'entrata in vigore di questi decreti delegati postula l'esigenza di un Consiglio superiore della magistratura ancora in fase di insediamento. Sostiene, quindi, che vi è la necessità di un intervento quanto più possibile tempestivo rivolto a sospendere l'efficacia dei tre decreti legislativi in modo che la loro effettiva operatività coincida con la costituzione dell'organo di governo in tutte le sue componenti, cosa che è già avvenuta da tempo (quindi, questa motivazione non è più valida). Stranamente,

Allora, anziché arrivare ad un atto di coraggio che la espone anche alla contestazione interna al Paese, cioè all'abrogazione *tout court* e alla presentazione in Parlamento di un disegno di legge che preveda tale abrogazione, ha deciso di adottare la politica dei piccoli passi del carciofo: si sospende immediatamente fino al mese di luglio dell'anno prossimo per poi abrogare definitivamente. Se lei avesse voluto modificare e accogliere l'appello del presidente Mancino

di norme già entrate in vigore senza creare alcun trauma all'interno del mondo giudiziario. Lei, signor Ministro, è sotto scacco dell'Associazione nazionale magistrati e ci è dispiaciuto leggere ieri dalle sue dichiarazioni proprio le frasi degli esponenti dell'Associazione nazionale magistrati!

per la cui decretazione d'urgenza mi risulta - lo crediamo tutti - che il Presidente della Repubblica abbia negato il proprio sigillo; tant'è vero che ci troviamo a discutere su un disegno di legge perché il Colle presumibilmente ha negato la propria firma su una decretazione d'urgenza che sospendesse l'entrata in vigore di una norma.

quale sarà l'atteggiamento di colui il quale, oggi seduto in quest'Aula del Parlamento, quando sedeva al Colle ebbe a ridire su alcuni aspetti di costituzionalità della norma tanto da rimandarlaal Parlamento per indurre le Camere correttamente a fare la propria parte, parte, introducendo modifiche che rendessero più costituzionale il testo. In quell'occasione il Presidente della Repubblica, che oggi siede in questo ramo del Parlamento, manifestò delle perplessità; successivamente il Parlamento si adeguò a quelle perplessità ed il Presidente della Repubblica promulgò quel testo. Vogliamo capire se oggi l'idea di quell'ex Presidente della Repubblica è cambiata o se è rimasto coerente a se stesso.

procedere. Se invece di dieci parla uno solo di voi ed indica l'irregolarità si può provvedere. Proclamo

Prego

Grazie,

parlare il senatore Divina.

della parola per argomentare sul tema che prima mi è stato impedito di illustrare. illustrare. Sono addirittura soddisfatto che il presidente Ciampi abbia votato contro tale questione pregiudiziale e che abbia assunto una precisa posizione politica su questo tema.

Mi domando se la necessità dei numeri imponesse anche questo sacrificio, soprattutto della sua immagine. Anche la volta il presidente Ciampi ha votato la fiducia al Governo non era più il Presidente di tutti gli italiani ma il Presidente della sinistra. Oggi, con questa sua presa di posizione pone anche qualche dubbio sulla sua correttezza istituzionale. Infatti, non si può intervenire prima approfittando dei propri poteri costituzionali e poi in sede politica. E' una commistione intollerabile.

registriamo un'altra triste giornata per le istituzioni del nostro Paese. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, io credo si sia detto molto valga la pena di ribadire quale è la natura vera del contendere. L'abbiamo fatto noi ed anche altri interlocutori che hanno parlato in questi giorni.

Quali sono gli effetti concreti e reali che questo provvedimento sta esplicando? Non è vero che il provvedimento è fatto, come ho sentito sostenere da qualcuno, da tre decreti legislativi che già, peraltro, sono intervenuti nella loro efficacia. Il provvedimento è formato da dieci provvedimenti legislativi diversi, alcuni dei quali pacificamente sono operativi da mesi e mesi; se la memoria non mi tradisce, il primo è diventato efficace addirittura a febbraio 2006. Credo che un Parlamento serio dovrebbe misurarsi su questo: è stata fatta una riforma importantissima, valutiamo serenamente quali sono stati gli effetti positivi e negativi. Non sono riuscito, né dal ministro Mastella,

dite qualcosa, come diceva un noto regista, entrate nel merito, nel concreto, senza ripetere continuamente che la riforma opera effetti devastanti: fatemi un che i procuratori siano soddisfatti, ad esempio, del decreto legislativo che cerca di rimettere un po' di ordine nel marasma di alcune procure, perché è noto a tutti che alcune grandi procure sono ingovernabili, dove il procuratore capo non sa nemmeno cosa fanno i sostituti; sono procure dove ogni sostituto va per la propria strada e poi le conseguenze le paga il Paese. Abbiamo avuto troppi esempi eclatanti,

in cui non ci sia un responsabile, un capo che governi: le uniche sono, o meglio erano, fortunatamente, le nostre procure. Oggi non è più così. Io non ho sentito una voce di un procuratore capo che denunciasse i guasti di questa riforma. Vorrei sentirli. Invece non è accaduto e addirittura un procuratore, lo cito per nome, il presidente Lepore, ha dichiarato

o il procuratore capo Lepore va immediatamente rimosso in quanto pericoloso sovversivo o incapace perché ha addirittura applicato, anticipando gli esiti della mia riforma, questi princìpi nella sua procura. Invece mi pare che

in* *deserto*, ovviamente non mi illudo che il mio appello venga ascoltato. Dovremmo avere un sussulto di dignità: vogliamo difendere la dignità del Parlamento, vogliamo stabilire il principio che è il Parlamento che legifera e poi tutti i cittadini, compresi i magistrati, obbediscono alle leggi? Non reagiamo più a nulla, abbiamo l'encefalogramma piatto. Si parla in questi giorni del fatto che il Parlamento non ha reagito agli insulti e alle minacce anche di morte che sono state fatte nei confronti del Papa e della nostra civiltà, ci soffermeremo

assolutamente fondata, perché evidentemente i suoi colleghi non lo perseguiranno mai - «tanto nessuno mi farà nulla perché tanto siamo noi che ce la cantiamo e ce la suoniamo, tanto siamo noi che decidiamo sulle questioni». Credo che questo sia un tema fondamentale; le leggi le fa il Parlamento o altri poteri? Come ricordavo l'altro giorno, questo è un tema che addirittura è mondiale. Avevo coniato anche un termine: la dicastocrazia, il potere dei giudici. Oggi si scrivono libri su questo tema,

Pochi giorni fa in Cassazione è stata completamente sovvertita una legge del Parlamento; si è detto «benissimo, il Parlamento ha fatto una legge sugli immigrati, ma noi decidiamo che così non va bene e la ribaltiamo completamente». Possibile che tutto questo venga accettato supinamente? C'è una cecità, credo, di una parte del Parlamento perché qualcuno per viltà, qualcuno perché c'è costretto in quanto è sotto ricatto, qualcuno per convinzione ideologica, è convinto che la classe dei magistrati possa essere utile all'azione di Governo e possa essere comunque utile averla al proprio fianco. È tuttavia una questione di democrazia; credo che non possiamo rinunciare al principio fondamentale per cui il potere è esercitato in nome del popolo, da chi il popolo ha eletto. È tutta qui la questione. Tra l'altro, da questo punto di vista, credo che alcune affermazioni del Ministro siano state anche abbastanza tragicomiche: il voler cancellare la targa che io ho voluto mettere nei tribunali. Ma, scusate, pensate all'eversione del ministro Castelli, che ha voluto che nei tribunali si scrivesse la prima frase che la nostra Costituzione per quanto riguarda la magistratura. Il Titolo IV, articolo 101, comma uno, dichiara: «La giustizia è amministrata in nome del popolo». Il ministro Castelli ha avuto l'ardire di fare affiggere

forse perché è timoroso di non riuscire a cancellare la legge e potrà dire «non sono riuscito a cancellare la legge, almeno la targa l'ho tolta». Evitiamo, per favore, queste cadute di stile, evitiamo queste prese di posizione così integraliste. Ripeto, rilancio l'appello, lo dico per l'ennesima volta - ma credo che mai come in questo caso *repetita* *iuvant* - che siamo disponibili a sederci attorno ad un tavolo

Siamo la patria di Galileo Galilei che ha fondato la scienza moderna, che ha rinunciato all'*ipse dixit* - a cui purtroppo tanta parte della nostra cultura è ancora agganciata per arrivare alla sperimentazione. Esaminiamo la realtà, sperimentiamo la realtà, verifichiamo cosa ci dice la realtà e sulla base di quei dati, che diventano oggettivi, ciascuno faccia le proprie proposte secondo la propria parte politica. Comprendo infatti perfettamente che sulla stessa realtà poi si possano giocare proposte diverse in funzione della propria ideologia, di come si vede la società, di quale si pensa debba essere il ruolo della magistratura nel nostro Paese.

di imbarazzante incertezza nel Senato, confermata da quanto accaduto oggi perché se sei senatori a vita non avessero votato la maggioranza sarebbe andata in minoranza, scrissi una lettera a tutti i senatori a vita dicendo che non derivando noi, se non per motivi storici, i nostri poteri dalla sovranità popolare, non potevamo interferire sui risultati del voto.

isolata, tant'è vero che sono dell'opinione che in una riforma costituzionale, se mai si farà, la figura dei senatori a vita debba essere abolita oppure limitata al diritto di parola e non al diritto di voto.

avesse avuto una esperienza tale da diventare Presidente della Repubblica. La Presidenza della Repubblica, salvo alcuni casi, è una vincita al lotto,

del Partito Socialista come Pertini, che era una bravissima persona, ma nel Partito Socialista non ha mai contato nulla, e come il sottoscritto, che nella Democrazia Cristiana non ha mai contato nulla, D'Alema ha un altro problema. Gli hanno messo due furbetti, uno del centro-destra e uno del centro-sinistra, e hanno detto: se va D'Alema siamo fregati perché Prodi dura per la vita.

vera vergogna - dissi: voi, cari magistrati se avete la sfortuna, leggetevi l'interrogatorio di Giovanni Falcone: una vergogna. Quando Giovanni Falcone fu chiamato davanti al Consiglio superiore della magistratura a discolparsi dalle accuse di Orlando Cascio fu una vergogna. Ho vomitato una volta solo in vita mia:

I senatori a vita scelti dai Presidenti della Repubblica per gli eccelsi meriti conquistati e i senatori che sono stati Presidenti della Repubblica e per ciò solo diventano senatori di diritto. Lo *status* di questi illustri colleghi è sempre stato oggetto di discussione serrata in Senato perché si ritiene che non appartengono alla stessa categoria democratica dei senatori eletti, ma appartengono pur sempre ai componenti del Senato e che, in quanto componenti del Senato, concorrono al *quorum* dei senatori ai fini dell'elezione del Presidente del Senato - e lo sappiamo - ma non concorrono al *quorum* se non presenti e votanti nelle sedute normali del Parlamento. Il Regolamento del Senato, in sostanza, ha già distinto dal punto di vista giuridico le due differenti categorie di senatori. Questo fatto di estrema rilevanza conforta le cose dette dal senatore Cossiga nel senso che è di tutta evidenza che i senatori di diritto e quelli a vita non possono, per ragioni di correttezza democratica, ma anche per ragioni di Regolamento parlamentare, modificare gli orientamenti politici presenti al Senato allorché si procede alle votazioni. Si tratta di un fatto di grande rilievo ed è evidente il motivo per il quale continueremo in questa legislatura ad assistere a fenomeni assolutamente sgradevoli dal punto di vista politico: senatori a vita che siano stati Presidenti della Repubblica e che, come tali, sono membri del Senato in quanto hanno rappresentato l'unità nazionale e in quanto non sono appartenuti ad una parte politica particolare, che improvvisamente al Senato diventano decisivi per gli equilibri politici. Ciò che è avvenuto poco fa nel voto sulla pregiudiziale è di enorme rilievo democratico perché il voto dei senatori a vita è stato determinante per la maggioranza politica, non è stato aggiuntivo rispetto ad esso. È stato determinante per il raggiungimento della maggioranza politica e addirittura per il *quorum*. Ma mentre per il *quorum* lo considero un fatto legato al Regolamento del Senato perché conseguenza del fatto che erano presenti e votanti, non è del tutto normale che concorrano alla formazione della maggioranza politica. Lo dico sia nei confronti dei senatori a vita che nei confronti dei senatori di diritto e invito a riflettere gli uni e gli altri su questo aspetto di estremo rilievo. In quest'Aula è di tutta evidenza che la loro presenza è graditissima, importante, dà dignità al Senato, ma non può modificare gli assetti politici che votando in Senato si determinano. Questo fatto è avvenuto stamattina in termini che suonano di insulto alla regola fondamentale della democrazia che si fonda sul voto dei cittadini e mi sembra molto grave che vi abbiano concorso senatori che siano stati Presidenti della Repubblica o che siano senatori a vita per decisione dei Presidenti della Repubblica, non in base al sorteggio, ma in base a meriti conquistati nel corso degli anni, che non sono meriti di elezione, altrimenti ovviamente sarebbero stati eletti. Non mi risulta che nessuno dei senatori a vita sia stato mai eletto al Senato, certamente non in questa tornata. Nessuno dei senatori di diritto è stato eletto al Senato. La regola dell'appartenenza al Senato non è quella della elezione, è un'altra ma non può modificare la naturale democraticità dei senatori presenti in Aula. Lo dico perché la materia tornerà Grazie, osannato da tutte le parti politiche per la sua integerrima, sovrana neutralità politica diventi determinante per una maggioranza politica anziché un'altra.

Cossiga siano formalmente inviate a tutti i senatori di diritto e a vita perché si rendano conto di cosa hanno fatto oggi, di cosa possono fare nel corso della legislatura; riflettano seriamente perché è una questione decisiva per la vita democratica del nostro Paese. Non è pensabile

il disegno di legge recante la cosiddetta riforma Castelli, che dava delega al Governo per molte parti, conteneva anche una norma che prevedeva l'abrogazione dell'ordinamento vigente.

può ovviamente riguardare la legge in vigore - ci mancherebbe altro - ma non può ripristinare norme abrogate a meno che non siano riproposte con un disegno di legge apposito che ne permetta il rientro in vigore. Per carità, si possono far rivivere tante cose per ragioni politiche anche dal punto di vista della Presidenza del Senato - ci possono essere persone in vita, non in vita - ma non si possono far rivivere norme giuridiche abrogate. Le questioni che allora pongo sono le seguenti.

Non c'è il rinvio a decreti legislativi che comportano l'abrogazione. L'abrogazione è oggetto che consegue a una parte della legge promossa dal ministro Castelli, che è diversa dai decreti legislativi.

suicidi nelle sentenze per farle annullare nel grado successivo, ma questo fa parte della vita giudiziaria. Il Parlamento non può, con proprie disposizioni legislative, far rivivere norme abrogate: questa è la questione. C'è una proposta del Governo che esattamente afferma

se si sospendono le norme in vigore, si fanno rivivere quelle vecchie e non interviene una nuova disciplina al 1° o al 31 luglio del 2007? Che cosa succederà se il Parlamento non emana una nuova disciplina?

dopo la sospensione non si farà più nulla, a meno che il Governo non ci dica che, anziché dar vita alle norme abrogate, rimangono in vigore, se non vi sarà la nuova legge, le norme dell'ordinamento Castelli. Allora il discorso